La seduta è aperta

*dal* *Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico:* «Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»

ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, d'intesa con i colleghi Russo Spena e Palermi, dichiaro che i Gruppi della Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani fanno proprio il disegno di legge n. 927, che mi vede primo firmatario, in materia di modifica della disciplina dei contratti a termine.

che si sono impegnati a "patinare" - come è stato riportato - di sola allegria la *kermesse* rispetto invece ai cori scanditi in particolare contro il Santo Padre,

il presidente Prodi promise: "Due terzi del tesoretto saranno destinati ad alleviare le situazioni di indigenti anziani e famiglie numerose". numerose". Signor Presidente, di questo tesoretto si parla tutti i giorni, dalle pagine dei giornali ai vari servizi... pratica ciò che si afferma in convegni di importanza nazionale ed internazionale e che poi viene regolarmente disatteso.

sull'inizio dell'esame della legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione italiana all'Unione Europea. Tale discussione assume particolare rilievo alla vigilia del Consiglio europeo del 21 giugno e delle decisioni che esso sarà chiamato ad assumere. In proposito, ho presentato una proposta di risoluzione, sottoscritta da altri 21 senatori. Vorrei richiamare la sua attenzione affinché l'Assemblea del Senato sia posta nelle condizioni di poter almeno avviare il dibattito prima della data del 21 giugno, in modo da dare il proprio contributo circa l'orientamento che il Governo italiano dovrà assumere in una riunione del Consiglio europeo che sarà, sotto ogni profilo, decisiva per il compimento dell'Unione Europea.

come prescrive il Regolamento, la presentazione di un disegno di legge di conversione in legge di un decreto‑legge. Ebbene, sono rimasto sconcertato nel sentire l'oggetto di tale disegno di legge: si tratta, infatti, di un decreto-legge

Signor Presidente, vorrei ricordare che già altri interventi, in precedenza, avevano richiamato la difficoltà della delegazione senatoriale a partecipare

Da quanto ne sapevo, fino ad oggi, la riformulazione - il famoso testo 2 - consisteva in piccole modifiche al testo che lo rendevano più chiaro e più comprensibile a tutti i colleghi, e a lei *in primis*. Ora, riguardo al decreto-legge sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, sono stati riformulati due emendamenti, uno all'articolo 8 e uno all'articolo 9.

ciò, le chiedo, signor Presidente, se questa può essere considerata una prassi consolidata, oppure se è un'eccezione che non fa la regola. Ripeto: se dobbiamo usare questi *escamotage*, cioè apporre la nostra firma all'emendamento per poi riformularlo, basta che ce lo dica e dal prossimo

presentare modifiche anche sostanziali e stravolgenti qualsiasi tipo di emendamento. PRESIDENTE. Credo che la presentazione di una riformulazione sia accettabile e possibile; starà poi alla Presidenza

noi dobbiamo valutare

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 giugno 2007. Come previsto dall'ordine del giorno, oggi pomeriggio riprenderà l'esame del decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania, con prosieguo e possibilmente conclusione nella giornata di domani. Anche a tal fine, la seduta pomeridiana di domani potrà protrarsi oltre il consueto orario. Il calendario di questa settimana comprende poi il seguito della delega sulla sicurezza sul lavoro e, ove possibile, il disegno di legge in materia di norme fiscali. Mercoledì 20 giugno, alle ore 12, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi i deputati. La chiama dei senatori dovrebbe avere inizio intorno alle ore 13,15, quindi dopo la conclusione della seduta antimeridiana. Martedì 26 giugno, alle ore 11, si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale sulla mozione Schifani ed altri sugli studi di settore. Nel pomeriggio, a partire delle ore 16,30, sempre di martedì, avranno luogo le dichiarazioni di voto e il voto su tale strumento ed altri eventualmente connessi. Il calendario della prossima settimana prevede poi, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, la legge comunitaria 2007, la delega per la liberalizzazione dei settori energia elettrica e gas e il disegno di legge collegato sul riordino dei servizi pubblici locali. Per la legge comunitaria si è proceduto, come previsto dal Regolamento, alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi, che potranno essere rivisti nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo. Il programma dei lavori è integrato con il disegno di legge sulla nomina elettiva dei giudici di pace, fatto proprio dal Gruppo della Lega, come provvedimento delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento.

recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti***

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a soli sette mesi di distanza dall'approvazione di un decreto-legge sulla stessa materia, sulla stessa situazione e con la stessa, anzi gravemente peggiorata, emergenza rifiuti, ci ritroviamo di nuovo in quest'Aula ad approvare un disegno di legge di conversione che non convince nessuno. Un altro decreto-legge da convertire che non ha spostato per nulla la grave condizione in cui è costretta la Campania. Con il precedente provvedimento il dottor Bertolaso, nella sua qualità di capo della Protezione civile, veniva nominato commissario per l'emergenza. Oggi Oggi esaminiamo questo provvedimento per ribadire che il dottor Bertolaso è commissario per l'emergenza rifiuti, solo con più ampi poteri. La verità è che, oggi come oggi, vi è una indiscussa e grave responsabilità dell'amministrazione regionale, che incassa, noncurante, l'ennesimo avviso di fallimento. In tutti questi anni, infatti, l'amministrazione regionale non è riuscita a superare l'emergenza, non ha avviato alcuna credibile forma di gestione dei rifiuti, non ha dato il via alla realizzazione degli impianti previsti per trattare i rifiuti. Ha lasciato insomma che il caos rifiuti crescesse a tal punto che ci vorranno molti anni per smaltire i milioni di tonnellate di spazzatura accumulata, mentre i cittadini campani hanno continuato a vivere in una situazione a dir poco offensiva per la dignità umana. Il decreto-legge ora all'esame costituisce una vera e propria denuncia dell'incapacità di gestire il problema rifiuti in Campania. L'emergenza non è un fatto temporaneo e contingente, ma ormai un fatto strutturale che, per essere risolto, ha bisogno di un vero e proprio mutamento di passo che porti alla responsabilizzazione di tutti gli attori, *in primis* degli enti pubblici territoriali. Tutto questo il decreto-legge n. 61 non lo fa o lo fa molto timidamente. Entrando nello specifico del testo, dobbiamo sottolineare come esso desti numerose perplessità. In particolare, sono molto discutibili le norme che individuano, senza alcuna previa consultazione con gli enti locali,

i siti delle discariche provinciali, scegliendo persino, in alcuni casi, parchi o aree naturalistiche. Il sito di Terzigno, all'interno del Parco del Vesuvio, è addirittura un sito nazionale di bonifica su cui sono stati già avviati interventi. Inoltre, l'articolo 2, al comma 1, prevede anche che si possono utilizzare come discariche provvisorie cave dismesse ed abbandonate, anche sottoposte a sequestro giudiziario. Oltre ad un'anomala sovrapposizione di ordinanze del potere legislativo e di quello giudiziario, si ricorda che le cave sequestrate, nella maggior parte dei casi, risultano molto spesso colme di rifiuti, anche pericolosi. Sarebbe quindi molto rischioso dal punto di vista ambientale aggiungere altri rifiuti in siti già compromessi. Non parliamo poi dell'articolo 7, che giudichiamo quantomeno improponibile per la parte che prevede la possibilità di aumentare per cinque anni l'importo della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per garantire la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Questo il trattamento riservato ai cittadini campani, che vedranno aumentare in maniera rilevantissima il tributo da pagare per un servizio che non ricevono o ricevono in maniera a dir poco discutibile. L'articolo 9 delinea il nuovo piano per il ciclo integrato dei rifiuti e riproduce alcuni articoli del decreto legislativo n.152 (Codice dell'ambiente), senza però assicurare tutte le garanzie di tutela dell'ambiente, di trasparenza, di tracciabilità dei rifiuti, così come si evince ed assicura il codice. Questo decreto ci fa comprendere come la strada da percorrere per superare l'emergenza rifiuti in Campania sia ancora lunga e travagliata. Non servono, per tornare alla normalità, gli *escamotages,* riproposti in questi giorni, di portare la spazzatura in altre Regioni o addirittura all'estero, in particolare in Romania, un Paese che già fatica a smaltire la propria correttamente. Dopo tredici anni di regime commissariale, in Campania la raccolta differenziata è ancora al palo, mentre si può dire che il 30 per cento di raccolta differenziata, e anche più, raggiunto in alcuni Comuni, dovrebbe far riflettere che se c'è una volontà politica ed amministrativa i risultati, effettivamente, si ottengono. Non esiste un piano per mancano ancora gli impianti di termovalorizzazione, impianti che chiudono il ciclo di smaltimento corretto dei rifiuti. I termovalorizzatori, che bruciano rifiuti e producono energia, presenti in quasi tutte le Regioni d'Italia, in Campania ancora non ci sono e se uno - quello di Acerra - sta per essere completato, lo si deve all'azione determinante del Governo di centro-destra.

Proprio l'emergenza rifiuti ha determinato un allarme sanitario in tutta la rete della Regione. Una ricerca commissionata dal Dipartimento della protezione civile ad esperti internazionali ha, infatti, evidenziato un aumento della mortalità in Campania da mettere in relazione allo smaltimento illegale dei rifiuti e alle discariche abusive. A Napoli e in tutta la Campania la crisi non è soltanto di natura igienico-sanitaria, ma anche e soprattutto istituzionale, perché in tali situazioni i cittadini non possono più avere fiducia nella Regione, nella Provincia e nel Comune. Allo stato, la popolazione esasperata ha preso l'iniziativa di rappresentarsi direttamente, occupando piazze, ferrovie e sedi istituzionali locali, oppure rivolgendosi direttamente al Capo dello Stato per avere garanzie e certezze, come hanno fatto a Parapoti o al comune di Quarto. Il comune di Ariano Irpino ha chiesto l'intervento del Senato per l'approvazione di un emendamento che garantisca, dando la massima certezza, che il conferimento dei rifiuti avvenga solo per venti giorni e che non possano essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino; il sito di Difesa Grande deve essere definitivamente chiuso. Ormai siamo alle ultime battute ed il testo che ora esaminiamo non è più quel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, perché è stato svuotato completamente della sua essenza; lo stesso commissario Bertolaso ha detto chiaramente che ora si procederà a rate e senza alcuna programmazione. Il consensoche potevamo dare al provvedimento era legato alla convinzione che fosse un passaggio necessario per tornare alla normalità. Trovarsi ora in Aula con l'emergenza ancora in corso ci dà pieno diritto di chiederci di cosa stiamo parlando. Ci troviamo in una situazione gravissima e pertanto abbiamo l'impressione che il meccanismo di solidarietà

*(AN)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento al nostro esame

si chiedono come mai in Campania non si riesca a risolvere una problematica che in ben tredici anni di emergenza si è trasformata, si è trasformata, come vediamo tutti i giorni dai servizi televisivi, in una vera e propria catastrofe. Proviamo quindi a fare chiarezza, con la speranza e l'auspicio che questo sia l'ultimo provvedimento e che si riesca a risolvere definitivamente questo annoso e spinoso problema. Innanzi tutto, voglio assicurare i colleghi che i cittadini della Campania, anche se sui giornali e nei servizi televisivi appaiono come un popolo in ribellione, non hanno alcuna responsabilità se non quella di avere dei rappresentanti istituzionali locali sui quali pesa tutta intera la responsabilità di una *mala gestio*. Queste mie affermazioni trovano sostegno nella stessa relazione del collega senatore Confalonieri, quando parla di errori istituzionali, di responsabilità degli enti locali e, in particolare, quando fa un chiaro riferimento al commissario straordinario Presidente della Regione Campania. Anzi, queste mie affermazioni trovano pieno riscontro anche nella relazione sulla Campania della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti della precedente legislatura. Lo scenario che descrive la Commissione nella sua relazione, soprattutto per gli anni 1999-2004, è infatti sconcertante. Il giro di soldi sperperati, signor Presidente, è spaventoso: si tratta di migliaia di milioni di euro sperperati tra spese generali, progetti, consulenze, convenzioni con professionisti, commissioni di gara, commissioni di collaudo. Sintomatico è l'esempio delle spese generali, che subiscono una lievitazione pazzesca: nel 1998 siamo a oltre 16.000 euro di spese generali; nel 1999 passiamo a 106.000 euro, che

in cui si è amministrata questa problematica e del motivo per cui si è poi incancrenita. Un riferimento va fatto anche alle tantissime società miste che si sono costituite solo per coprire poltrone, per dare incarichi, con consigli di amministrazione sempre composti di sette o otto persone, con revisori dei conti e consulenti. La Campania è già una Regione notissima

Emblematica è la vicenda sulla società mista PAN: in Campania era così importante, signor Presidente, costituire una società che avesse il compito di installare un *call* *center* per informare i cittadini sul disagio ambientale e su quello dei rifiuti? l'attività del commissariato dal 1999 al 2004 è stata concentrata solo sulla gestione dell'emergenza e non sul programmare il superamento dell'emergenza. Questo è scritto, in sintesi, nella relazione finale della competente Commissione di inchiesta e sono qui ipotizzate tutte le responsabilità. Intanto, i rifiuti continuano a girare in Campania, facendo la felicità, signor Presidente, delle organizzazioni criminali.

«La criminalità organizzata» - dichiara il prefetto Catenacci il 15 marzo 2005 - «sorride per l'andamento odierno della situazione in Campania; infatti, sono aumentati i trasporti ed il ritardo della costruzione delle discariche e dei siti di smaltimento determina l'aumento dei viaggi in direzione di altre località. Le indagini delle forze di polizia e della magistratura rilevano sospetti di collusione o di condizionamento tra imprese di trasporto e criminalità organizzata». quindi leggere i risultati della Commissione parlamentare di inchiesta; lì sono indicate tutte le responsabilità. osservare le cose che ha lasciato scritta la Commissione per vedere come risolvere il problema. Se si aggiunge che nulla è stato fatto, né si sta facendo, per incentivare la raccolta differenziata e per gli interventi di bonifica ambientale, allora si comprende veramente e seriamente il disagio il disagio e l'esasperazione dei cittadini della Regione Campania. Va ricordato che in Campania sono stati individuati moltissimi siti di cui alla legge n. 426 del in quella Regione c'è un'anomalia tutta campana: c'è un commissario per l'emergenza rifiuti, il dottor Bertolaso,

sia noto a tutti il disagio ambientale e che gli interventi di bonifica non sono stati fatti, rimane ancora lì imperterrito e senza timore di alcuno. Non ha timore di alcuno: continua imperterrito a rivestire la carica di commissario

solitaria, disposizioni ai vari Governi che si sono succeduti. Veda, signor Presidente, abbiamo a cuore le sorti della nostra Regione e in tal senso ci siamo posti con spirito costruttivo. Con l'altro provvedimento indicammo una strada, quella di individuare i Presidenti delle Province, affinché si assumessero una responsabilità.

i Presidenti delle Province? Siamo contenti che in questo provvedimento, per esempio, sia stata raccolta una nostra preoccupazione, chiediamo però all'Aula anche di dare un messaggio a fronte di un altro emendamento che abbiamo presentato e che riguarda la tariffa che i cittadini pagano. I cittadini sono vessati da un servizio che non ricevono e da una tariffa che è aumentata in maniera vertiginosa.

l'UDC è particolarmente impegnata su questa vicenda per un insieme di ragioni. Il Gruppo UDC voterà contro la conversione in legge di questo decreto-legge perché sostanzialmente lo riteniamo non soltanto fortemente incostituzionale - e di ma radicalmente inutile rispetto a quanto avvenuto fino ad ora in Campania. Ho ritenuto necessario, prima dell'intervento oggi al Senato,

molto stancamente, ha approvato un ordine del giorno molto lungo, che spiega perché noi votiamo contro questo decreto‑legge. Questa maggioranza ha avuto anche

il senso dell'ordine del giorno di Napoli - di chiedere al Governo, nell'ultimo punto dell'ordine del giorno, di abrogare gli articoli 7 e 8 di questo decreto-legge, prevedono che il gigantesco costo aggiuntivo per far finta di completare lo smaltimento dei rifiuti venga sopportato dai cittadini della Campania:

Il Governo cioè prende atto della propria incapacità di far fronte ai problemi dell'emergenza, prende atto del fatto che non vi è stata la risposta ai problemi dell'emergenza da parte degli enti locali della Campania, e chi fa responsabile del pagamento? I cittadini della Campania. Quando poi si parla della gente che reagisce, insulta e grida e si dice che questo è contro la democrazia, ci si rende conto che questo decreto è un continuo è un continuo incitamento alla reazione popolare contro questo Governo e contro le amministrazioni regionali e locali della Campania? Questo è un decreto‑legge che suona insulto alle popolazioni della Campania. Fanno bene a dire che il Governo se ne deve andare il più presto possibile. Occorre capire che non è un problema della Campania, legato a un fatto quasi antropologico dei campani rispetto al problema dell'immondizia: è un problema del Governo della Repubblica, del Presidente della Regione Campania e dei Sindaci, in particolare di Napoli, rispetto a questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi non avrebbe risolto i problemi dello smaltimento, ma sarebbe stata almeno un gesto comprensibile di responsabilità politica e amministrativa. Vorrei allora avanzare una richiesta al relatore, se mi fa la cortesia di ascoltare.

chieda formalmente lui l'abrogazione degli articoli 7 e 8 di questo decreto-legge; chieda cioè che i cittadini della Campania non siano chiamati essi stessi a far fronte alle spese di questo fantomatico

questo decreto non può rimanere tale perché è contro il principio fondamentale in base al quale si paga a fronte di servizi resi, non a fronte di servizi non resi. La TARSU è un'imposta, un tributo, una tassa (a seconda dei criteri che si vogliono usare) da corrispondere a fronte di un minimo ragionevole smaltimento dei rifiuti. Ma se questo non è avvenuto, a fronte di che cosa i cittadini dovrebbero pagare questo di più? Ci si rende conto che si chiede una cosa impossibile?

dev'essere tale da garantire le spese aggiuntive. Cioè, non sappiamo neanche di che entità è: una cosa mostruosa! I cittadini della Campania dovrebbero essere chiamati a pagare cifre pazzesche per un risanamento che non è stato realizzato. Inoltre, questo decreto contiene un altro fatto istituzionale molto preciso (lo dico al Presidente del Senato perché se ne faccia carico, anche se capisco che il Presidente del Senato non può entrare nel merito degli atti legislativi). In questo decreto-legge vi è un articolo, il 2, che contiene una previsione di tecnica eversiva costituzionale. in esso vi si afferma (credo per la prima volta nella storia repubblicana, non so se vi siano precedenti) che un provvedimento giurisdizionale di sequestro di una discarica può essere posto nel nulla dall'autorità amministrativa.

di presentare un proprio, volontario emendamento nel quale si impedisca di dire che l'autorità amministrativa può superare il sequestro della discarica. Non è una questione generica; quando, qualche giorno fa qualcuno ha chiesto cosa stanno facendo ad Ariano Irpino: ebbene, stanno facendo una cosa dovuta anche a questo decreto, perché la discarica di Ariano Irpino era chiusa per provvedimento giurisdizionale esecutivo stata riaperta per volontà dall'autorità amministrativa. Mi sembra che, rispetto agli atti di eversione costituzionale, l'unica tutela sia quella di impedire una violazione della Costituzione così clamorosa. Non lo dico per legittimare la protesta degli amici di Ariano, ma per far capire che li avete portati all'esasperazione politica e costituzionale. Non è mai avvenuto in questo Paese che si sia immaginato di porre una questione del genere! Chiedo quindi formalmente che l'articolo 2 di questo decreto-legge, che espressamente prevede che il commissario delegato, in questo caso Bertolaso ma un commissario delegato in generale, possa disattendere anche l'ordine dall'autorità giudiziaria, che quindi viene messo da parte, cioè viene cancellato. Così come prima chiedevo e chiedo, a nome all'UDC, che non siano i cittadini della Campania a pagare per questo disastro, ora chiedo che l'autorità amministrativa, fosse anche quella del Governo Prodi (che tutti sappiamo essere quasi divina, dotata di poteri straordinari), non possa disattendere provvedimenti giurisdizionali.

contro Berlusconi ogni cosa sarebbe consentita. No: questa cosa è stata fatta contro i cittadini dalla Campania, contro i magistrati, anche quelli che hanno deciso che dev'essere chiusa una discarica perché esiste il sospetto di infiltrazioni camorristiche. Che cosa dobbiamo pensare

che in Campania da questa vicenda drammatica si possa cominciare ad avere un minimo di speranza di uscita? Dopo questo chiedo: ma è la prima volta che si interviene? Sembra quasi che fino ad ora siamo stati inerti. Non Non molto tempo fa chiedevo al collega Libè, che con estrema solerzia si sta occupando dell'insieme della vicenda ambientalista posta in essere da questo decreto: quando abbiamo approvato un altro decreto-legge che dava poteri straordinari e, sembrava, risolutivi,

Dobbiamo fare un nuovo decreto-legge per legittimare l'incapacità del Governo a fare ciò cui doveva provvedere prima? Noi siamo, quindi, contro la finzione della non reiterazione di un decreto, perché di questo si tratta, dal momento che i poteri erano già stati dati e non sono stati esercitati.

che siano formalmente cancellati gli articoli che prevedono che i cittadini paghino per questa iniziativa del Governo e che non si consenta che l'autorità amministrativa venga posta in vantaggio rispetto all'autorità giurisdizionale. Ma vi è un ultimo punto, che mi sta molto a cuore. Questo decreto-legge sembrava quasi volere in qualche misura individuare finalmente per autorità i luoghi della discarica: ebbene sì, decidiamo noi dove c'è la discarica e come la

Ad un Governo che dopo tanti anni non è riuscito a far nulla, al riguardo, e che fa credere ai cittadini una cosa del genere? Dunque: Serre non c'è, Terzigno è una presa in giro, di Ariano Irpino abbiamo detto, vi è un'autorità amministrativa che supera quella giurisdizionale. Onestamente, non conosco personalmente Sant'Arcangelo Trimonte in Provincia di Benevento. Ritengo che, da questo punto di vista, essendo l'ultima delle località della Campania, non possa essere quella che subisce il divieto generalizzato di discarica in tutto il resto della Campania. La domanda è quindi la seguente: siete stati in grado di proporre delle alternative?

piccolo comprensorio. Questa sarebbe l'alternativa reale, credibile, che la gente tollererebbe. La gente di quattro o cinque Comuni provvede alla discarica che riguarda quegli stessi Comuni, non certo l'intera Regione Campania. Volete capire, una volta per tutte, che questa pretesa di autorità nazionale

Grazie,

su questo argomento. Un commissariamento che dura dal febbraio 1994 e passato attraverso commissari prefetti, Presidenti della Regione, di nuovo prefetti, fino ad arrivare

in pochi minuti - ricordare le tappe che hanno portato all'emergenza di questi giorni. In un bando di gara del 1998 si ipotizzava che l'aggiudicatario della gara, il gestore unico, avrebbe dovuto occuparsi dell'intera filiera dello smaltimento dei rifiuti. L'impianto della

comunque ci si voglia rivolgere alle tecnologie più innovative, comporta degli impatti sull'ambiente. Ripeto, prevedere che chi si aggiudica la gara sceglie i luoghi è il primo errore,

a proprie spese fuori da quella Regione negli impianti a ciò destinati. Siccome l'emergenza crea emergenza e con i poteri commissariali straordinari si può derogare alle norme, come avviene anche in questo decreto, con un'ordinanza - una delle molteplici emanate

Nel 1998 si era deciso di chiudere le discariche perché c'era un piano industriale, che prevedeva impianti di CDR e inceneritori; nel frattempo, invece, le discariche non sono state chiuse

e dobbiamo saperlo nel momento in cui andiamo a votare il decreto - che ad ottobre o a novembre, quando entrerà in funzione la prima linea dell'inceneritore, in Regione Campania

e stiamo continuando a produrre un combustibile non a norma, che continuiamo stoccare in aree che consumano ogni mese 40.000 metri quadri. In tutto ciò, è di oggi la notizia che si apre finalmente la discarica di Ariano Irpino

all'uso delle aree protette: a Terzigno, nel Parco del Vesuvio, si andrà solo per una ricomposizione morfologica, per chiudere alcune cave che sono state negli anni sversatori della camorra e per dire che lì possiamo compiere un'operazione importante, portandoci una frazione organica,

il danno prodotto dall'articolo così com'era stato scritto. Così come interveniamo sull'esigenza di un piano, dato che non si può scrivere in un decreto che si fa un piano industriale: dobbiamo comunque rispettare la legge, le normative nazionali ed europee, per cui diciamo che il piano deve essere effettuato, ma deve essere un piano di ciclo integrato dei rifiuti e su questo abbiamo lavorato e bisognerà chiederemo - che ogni mese il commissario Bertolaso riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione, per evitare di trovarci alla scadenza, a dicembre, di nuovo in una situazione di emergenza, con i rifiuti per strada e il Parlamento ad occuparsi di questo. osservazioni che riguardano la tariffa. Riteniamo che il costo dell'emergenza non possa essere pagato dai cittadini e che, così come avviene in altre Regioni d'Italia, i cittadini debbano pagare e i Comuni debbano applicare tariffe e tasse che devono coprire il costo dello smaltimento, ma pensiamo che i cittadini e i Comuni debbano pagare esclusivamente il costo ordinario, ossia

alcune proposte emendative che saranno sottoposte alla discussione e all'attenzione dell'Aula. Questo pensiamo che sia corretto anche nei confronti di alcune sollecitazioni che venivano da colleghi della Lega Nord: non si afferma che l'emergenza campana debba andare a carico di altre Regioni o altri cittadini,

Di queste, ogni giorno ne restano 3.500 come ecoballe e 2.300 come FOS. Tutto ciò va stoccato, va in discarica.

pensiamo di fornire due risposte: quella all'emergenza, senza quindi mettere piombo sulle ali del commissario Bertolaso, e nello stesso tempo quella di dare garanzie per la tutela dell'ambiente, la salute dei cittadini, la salvaguardia delle aree protette, la salvaguardia dell'autonomia e dei poteri di altri organi dello Stato e delle autonomie locali.

sarei tentato di chiedere di poterlo fare mio e riproporlo integralmente a quest'Assemblea. Sarebbe peraltro un peccato di pigrizia

Sodano. Proprio partendo dall'aspetto dei dati, che forse sfugge esattamente all'attenzione di questa Assemblea, credo sia opportuno illuminare cosa sta accadendo ed è accaduto in Campania: vi sono circa sette milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti non smaltiti; vi è un territorio che viene divorato quotidianamente nella misura di circa 40.000 metri quadrati al giorno per il deposito delle ecoballe; vi è una produzione giornaliera di circa 7.500 tonnellate di rifiuti, di cui solo una minima parte rientra nel ciclo della raccolta differenziata, perché la restante e prevalente parte, sia pure

la Regione Campania e chi l'amministra. Purtroppo, ancora una volta il Parlamento è costretto a prendere atto del totale fallimento della politica di trattamento e smaltimento dei rifiuti da parte della Regione Campania,

sulla più iniqua delle sanzioni. Ai cittadini campani, che vivono realmente in una condizione che è al di sotto di quello che è il minimo di dignità che qualunque comunità deve assicurare ai propri figli, si vuole oggi addirittura imporre di farsi carico di farsi carico delle vergognose inefficienze che hanno caratterizzato la politica della regione Campania negli ultimi anni, caricando sulla tariffa il costo teorico perché tanto teoria rimane, perché in pratica questo provvedimento (e traspariva addirittura dalle accurate preoccupazioni del presidente Sodano) non risolverà assolutamente nulla, perché non ci sono i tempi e non ci sono gli impianti e ci troviamo a fare una copia a carta carbone di un provvedimento già preso sette mesi fa e che ha dimostrato di per sé, proprio in relazione a quella assoluta mancanza di una politica regionale di smaltimento dei rifiuti, di essere completamente fallimentare. Nel contesto di questo ragionamento, che è sì politico da un lato, ma è parimenti operativo dall'altro, non possiamo non tornare per un attimo, signor Presidente, onorevoli colleghi, su tre punti che sono stati mirabilmente trattati - ripeto - in quell'intervento che certamente vorrei fare mio, anche perché certamente espresso con ben altre parole. Il primo è relativo a questa sorta di peccato mortale che dal punto di vista giurisdizionale andiamo a compiere nel momento stesso in cui si prevede addirittura di sostituirsi a quello che è il legittimo potere esercitato dalla magistratura nell'adempimento delle proprie funzioni, addirittura in relazione a discariche che sono oggetto di provvedimenti giudiziari legittimamente adottati nel corso di indagini tuttora pendenti, con tutto quello che è il corollario che ne discende, in una società già profondamente degradata e inquinata dalle interrelazioni esistenti fra criminalità organizzata e ciclo di smaltimento dei rifiuti. Il secondo è legato all'obbligo, e non alla semplice facoltà, per i Comuni della Regione Campania - e certo su un Comune in particolare e su come è stato amministrato proprio in relazione allo smaltimento dei rifiuti (mi riferisco ovviamente alla città capoluogo di Regione) molto si potrebbe dire, tenuto conto che tra l'altro è la principale produttrice di questi rifiuti non smaltiti - di avvalersi necessariamente, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania del 10 febbraio 1993, che sappiamo perfettamente non avere funzionato, e che quindi come non hanno funzionato nel passato, non funzioneranno nel presente e non funzioneranno nel futuro.

le mende profonde che caratterizzano questo provvedimento, che bene sono state delineate in questo concetto di oscenità costituzionale e parlamentare, ma appunto la più iniqua delle previsioni è giusto che in quest'Aula risuoni ancora una volta come memento a tutti noi, lo stesso presidente Sodano ha avuto il coraggio, glie ne do atto, di ricordarla al Governo (un Governo che in Commissione, è bene dirlo, colleghi, è stato sordo a qualunque proposta emendativa che non fosse assolutamente di dettaglio e che dobbiamo presumere che anche in Aula avrà lo stesso atteggiamento) ovverosia, ripeto, il fatto che gravissime responsabilità altrui, che hanno abbassato la soglia della qualità della vita in Campania al di sotto di un qualsivoglia livello di accettabilità, debbano nuovamente essere pagate dai cittadini campani. Il Gruppo di Alleanza Nazionale questa oscenità non la consentirà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustri rappresentanti del Governo, dopo meno di un anno dall'ultimo decreto-legge sull'emergenza dei rifiuti, siamo chiamati ancora una volta ad affrontare la gravissima crisi che attanaglia la Regione Campania. La situazione attuale, com'è noto, ha assunto dimensioni ancora più allarmanti di quelle che indussero il commissario Bertolaso, in occasione del precedente decreto, ad equipararla ad una vera e propria calamità naturale. Per la verità, nell'ottobre dell'anno scorso in molti avevamo confidato che gli strumenti e i poteri messi a disposizione del commissario potessero consentire il superamento delle criticità connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti e l'avvio di un percorso virtuoso, fondato su una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, su un'opera di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, su un significativo aumento della raccolta differenziata, sulla realizzazione di impianti di compostaggio, sulla messa a norma degli impianti di CDR e sull'attivazione di almeno un termovalorizzatore. Addirittura da alcuni molto ottimisticamente si ritenne che quello dell'ottobre 2006 sarebbe stato l'ultimo provvedimento con il carattere dell'urgenza su tale materia. Dovremmo forse indagare, cari colleghi, le ragioni che hanno impedito a quella normativa, nella quale veniva riposta tanta fiducia, di conseguire gli obiettivi fissati. Mi limito ad osservare che in quel decreto era prevista l'apertura di tre discariche per fronteggiare l'emergenza, mentre invece ne fu aperta una sola, quella di Villaricca, che fino alla fine del maggio scorso ha funzionato come unica discarica per i rifiuti di tutta la Regione Campania. Probabilmente, se non fosse stato modificato il piano originario del commissario, oggi non ci troveremmo di fronte all'acuirsi dell'emergenza che sembra non avere mai fine e che il Capo dello Stato non ha esitato a definire tragica. Di fronte a questo fallimento, molti si ergono a censori e giudici, pronunciando giudizi e addebitando responsabilità. Io non intendo iscrivermi né al partito dei difensori d'ufficio né a quello degli acritici accusatori. Ritengo però che dovremmo tutti evitare strumentalizzazioni politiche e atteggiamenti di sciacallaggio, nella consapevolezza che della gestione dell'emergenza si sono occupati tre presidenti della Regione in qualità di commissari di diversa estrazione politica, Rastrelli, Losco e Bassolino, e che quest'ultimo da ormai tre anni è stato sostituito da due alti funzionari dello Stato: prima il prefetto Catenacci ed attualmente il capo della Protezione civile, dottor Guido Bertolaso. È anche opportuno sottolineare che se indubbiamente le maggiori responsabilità vanno ascritte a livello regionale, esistono competenze e funzioni anche in capo al Governo nazionale. E qui devo dare atto al presidente Matteoli di avere affermato, in occasione della conversione del precedente decreto, che sia il Governo di centro-sinistra sia quello di centro-destra che hanno attraversato questo decennio non hanno trovato una soluzione e quindi possono avere responsabilità. In tale quadro credo che le condotte e le scelte poste in essere in questi lunghi anni debbono essere vagliate in maniera molto più approfondita e in sedi più appropriate, quale la Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, tenendo anche conto del fatto che la magistratura ha avviato numerose inchieste dalle quali potranno - io lo spero - venire risposte chiare anche con riferimento al ruolo della criminalità organizzata. Venendo al disegno di legge al nostro esame, non entro nel merito analitico delle norme, riportandomi alle valutazioni espresse dal relatore in ordine all'impianto complessivo del provvedimento e alle specifiche misure che sono state introdotte. Posso solo ribadire nella sua situazione in cui versa la Campania non vi sono allo stato alternative possibili; occorre dare massima fiducia al commissario e confidare nei provvedimenti che il decreto gli consente di attuare. qualche breve considerazione sull'articolo 3, che prevede il divieto di localizzare nuovi siti di smaltimento finale dei rifiuti nel territorio dell'area flegrea, ricompresa nei comuni di Giugliano, Villaricca, Qualiano e Quarto, divieto che in Commissione è stato esteso anche alle aree protette ed ai siti di bonifica di interesse nazionale. Lo faccio solo per perché da taluni è stato avanzata qualche perplessità su tale disposizione e da alcuni senatori di Forza Italia se ne è proposta addirittura la soppressione. Certamente non si tratta di una scelta casuale o irrazionale, in quanto trova fondamento in fatti inoppugnabili che non hanno destato particolare clamore solo perché le proteste dei cittadini hanno assunto forme non molto eclatanti, e anche per il grande senso di responsabilità e la compostezza istituzionale degli amministratori dell'area giuglianese, i quali però non sono più disposti ad accettare altre azioni devastatrici del territorio e pericolose per la salute pubblica. Provo a ricordarli i fatti che hanno ispirato l'articolo 3 del decreto, poiché credo che qui molti non li conoscano. Il traffico dei rifiuti speciali che, da ogni parte d'Europa, in particolare dal Nord Italia, sono stati trasferiti nel triangolo Giugliano-Villaricca-Qualiano;

la discarica di Masseria del Pozzo nella quale, per alcuni anni, sono stati depositati tutti i rifiuti della città di Napoli, nell'ordine di 4 milioni di metri cubi invasati; la discarica Novambiente, la discarica Cava Giuliani e la discarica Schiavi, tutte ricadenti nell'area giuglianese, nell'ordine complessivo di 3 milioni di tonnellate. I fatti sono anche l'ordinanza del commissario di Governo che, nel 2004, dispose l'apertura della discarica di Settecainati, ai confini tra Giugliano e Qualiano - sempre lì! nella quale è stato stoccato circa un milione di tonnellate di rifiuti, nonché l'ordinanza commissariale del 10 giugno 2006, con la quale si dispose l'utilizzo della cava Masseria Riconta, nel comune di Villaricca, che ha assorbito oltre mezzo milione di tonnellate di rifiuti per fronteggiare, non l'emergenza di quell'area, ma di tutto il territorio regionale. I fatti sono un impianto di CDR tra Giugliano e Qualiano, con annesso piazzale ove sono stoccate 400.000 ecoballe. I fatti sono lo spettacolo agghiacciante che si presenta a Taverna del Re, nel comune di Giugliano, dove è accatastata una quantità gigantesca di ecoballe e dove si procede ancora, a ritmi forsennati, a divorare i rigogliosi frutteti dei terreni circostanti per realizzare nuove piazzole di cemento ove stoccare il falso combustibile che esce dai CDR nell'ordine di ben 2.200 ecoballe al giorno. Lo ha ricordato il presidente Sodano, lo hanno ricordato anche colleghi che mi hanno preceduto. E io su questo ho presentato un ordine del giorno per fissare un limite temporale entro il quale far cessare questa attività di saccheggio ulteriore del territorio. I fatti, infine, sono le indagini del Consiglio nazionale delle ricerche, che, nella relazione del giugno di quest'anno per la Commissione ambiente della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze ambientali provocate dallo smaltimento dei rifiuti, a proposito della Campania evidenzia gli aumenti significativi della mortalità per numerose forme di neoplasia, nonché delle malattie circolatorie e del diabete - guarda caso, guarda caso! - nei Comuni di Giugliano, Qualiano e Villaricca, aree in cui erano stati censiti ben 39 siti di smaltimento dei rifiuti, la maggior parte contenenti rifiuti pericolosi. Con riferimento a tale dato epidemiologico, ha ragione il collega Piglionica quando afferma che bisogna evitare di spargere terrore attraverso allarmismi immotivati, in quanto l'incremento di tumori e di altre patologie è correlato prevalentemente allo sversamento illegale di rifiuti tossici, che ha visto saldare gli interessi di imprenditori senza scrupoli, soprattutto del Nord, con quelli criminali della camorra locale. Se questo è vero in un contesto ambientale normale, nel quale l'inquinamento prodotto da una discarica controllata non determina effetti particolarmente dannosi alla salute, non lo è invece per un contesto completamente devastato, quello di cui all'articolo 3, gravato, da oltre un decennio, da decine di discariche, legali e abusive, che non è quindi più in grado di assorbire anche il benché minimo incremento di agenti inquinanti. In queste aree, e su questo so che il collega Piglionica è d'accordo, l'unica cosa da fare è bonificare, non certo aprire nuove discariche. Questo è il principale dovere che abbiamo nei confronti di una comunità che ha visto oltraggiato e deturpato il proprio paesaggio naturale, fatto di bellissime e fertili campagne, comunità alla quale il bisogna restituire fiducia nel futuro. E qui, concludendo, tornano attuali le parole pronunciate da Carlo Levi in un memorabile discorso in quest'Aula del Senato: «il paesaggio italiano che noi vogliamo difendere» - disse Levi - «non è un bene estetico che stia fuori dalla storia. Il paesaggio italiano non è altro che la storia vivente del popolo italiano. Il paesaggio non è che l'uomo, la campagna, non è che il contadino, le infinite generazioni di contadini che l'hanno lavorata e costruita come un'opera d'arte». Un luogo quindi non è solo il suo paesaggio, ma, replicando ancora le parole di Levi: «la sua stessa esistenza storica e la sua capacità di futuro». Non distruggiamo questa speranza di futuro, sostenendo la esclusione contenuta nell'articolo 3,

soleva spesso dire Einstein che i problemi non possono essere risolti con la stessa cultura che li ha prodotti. Credo che questa citazione ben si adatti alla situazione

citando non solo una incapacità generale che ha prodotto errori su errori ma su cui - come ha giustamente fatto riferimento il collega Palumbo - si è inserita pienamente, lucrando - la chiamiamo ecomafia - la camorra, la criminalità organizzata, che ha fatto sì che in Campania vi siano più di 600 discariche

di poter continuare per questa strada, stiamo sbagliando ancora una volta e ce ne dovremo assumere la responsabilità anche come Parlamento. Per questo motivo la Commissione è intervenuta su alcuni profili molto delicati di questo decreto,

Guardate! Se si pensa che ancora una volta si tratti di un altro piano industriale per qualche altra impiantistica da localizzare - non so - tra una rivolta e l'altra, credo non sia quella la strada giusta: significa che bisogna agire, come si è proceduto in altre Regioni, con serietà e serenità, ridando fiducia ai cittadini anche sulla raccolta differenziata. Su questo insisteremo fino alla fine: bene ha fatto la Commissione ad inserire questi punti. Questo decreto, Presidente, provoca sofferenza in molti di noi in molti di noi ed abbiamo lavorato con la collaborazione di tutti per cercare di ridurre il danno e per dare uno strumento che possa farci uscire dall'emergenza. Ricordiamoci, dall'emergenza si potrà uscire seriamente rinnovando il rapporto con i cittadini solo se alla fine disporremo di questo benedetto Piano regionale dei rifiuti, gestito con razionalità e serietà.

vorrei fare una replica molto sobria, perché ho ascoltato un dibattito dai toni a volte aspri, che però ripercorre la storia drammatica di questa situazione. Esso ha evidenziato, in termini anche trasversali, sofferenze, letture ed analisi che sono anche condivisibili. È un dibattito che ha ripetuto in questa Aula una discussione seria che abbiamo svolto in Commissione.

in questo momento a noi tocca fare una scelta, una scelta che individui una priorità.

se questo decreto sia perfetto ma la seguente: se oggi non convertissimo in legge questo decreto faremmo un favore alla Campania? Faremmo un favore ai cittadini della Campania? Faremmo un favore a quella terra oppure creeremmo un'aggiunta, un'addizionale, un *surplus* di pesantezza? Mi sembra perfino una domanda retorica.

di convertire in legge un decreto-legge, che non è certamente il provvedimento migliore che potrebbe esserci ma che va nella direzione indicata in molti degli interventi che ho sentito, oppure non solo non faremo un grande favore alla Campania ma creeremmo una situazione insostenibile.

non è figlio di una congiuntura astrale particolarmente sfavorevole ma evidenzia responsabilità precise, che in questo periodo di tempo hanno visto all'opera diverse situazioni: sei commissari. È del tutto evidente che queste responsabilità vanno interrogate ma occorre anche una grande assunzione di responsabilità. Ognuno può legittimamente scegliere di indicare una priorità piuttosto che un'altra ma è del tutto evidente che oggi siamo in questa situazione, lo dicevo anche nella mia relazione introduttiva, per

delegato, rinnovandoli, dei poteri che consentono di intervenire sull'oggi, in termini di individuazione di quattro discariche e in termini di individuazione di poteri in questa direzione, è un dovere che il Senato non può non prendere in considerazione. Ma ciò è correlato (lo ricordavano molte senatrici e molti senatori) ad un altro punto: se davvero vogliamo, e tutti ce lo auguriamo, che questo sia l'ultimo decreto sull'emergenza, va da sé che che nell'arco di questi mesi occorre arrivare a definire un piano ordinario per un ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti in Campania. Nel decreto

non può diventare un altro pio desiderio, perché di pii desideri credo siano lastricate le strade della Campania e dell'Italia: una volta tanto, dobbiamo portare a casa un risultato e a me pare che sommessamente, senza grandi enfasi, in questo decreto la combinazione, l'interrelazione, il combinato disposto, tra i

di questa valenza, essi sono stati costruiti anche in una relazione positiva con il Governo. L'ultimo di questi emendamenti è di stamane: una relazione virtuosa tra la Commissione

l'emendamento 1.500, che vincola le deroghe all'emergenza in maniera chiara, e l'emendamento 1.19, che parla di Terzigno. Sappiamo tutti dov'è Terzigno, sappiamo tutti che cos'è, però l'emendamento parla di Terzigno come discarica cui afferire alcuni rifiuti particolari e precisi, non tutto il possibile. Ricordo poi l'emendamento 2.22, che fa riferimento a quanto sentito anche in quest'Aula, in una combinazione che mette in equilibrio la necessità del commissario di utilizzare anche siti sotto sequestro con le prerogative della magistratura per il futuro.

all'articolo 3. È un emendamento che ho presentato come relatore, figlio di un accordo che è stato fatto nella Commissione con i commissari presenti e con il Governo, in relazione con i livelli istituzionali e le istituzioni democratiche di Irpino. Questo emendamento consente di poter gestire l'ordinanza che il Governo ha adottato non più tardi di qualche giorno fa.

Signor Presidente, il decreto‑legge di cui proponiamo la conversione qui al Senato fotografa la situazione di grave emergenza e di perdurante difficoltà che attraversa lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

che individuava come commissario delegato per l'emergenza il capo del Dipartimento della protezione civile, proprio come risposta alla gravità della situazione che si era venuta nel frattempo a determinare. Questo nuovo decreto si è reso necessario proprio per dotare il commissario delegato di strumenti di intervento e operativi che evidentemente non era possibile apprestare con il semplice ricorso al meccanismo delle ordinanze della Protezione civile. Questa sottolineatura di partenza, che deve rappresentare un elemento di piena consapevolezza da parte dell'Aula del Senato, giustifica pure la previsione normativa di interventi ai limiti della legislazione ordinaria. D'altra parte, se non fosse stato necessario ricorrere a strumenti eccezionali, di copertura anche giuridica per gli interventi del commissario, non sarebbe stato nemmeno necessario il ricorso al decreto‑legge in questione. Desidero ringraziare in particolare i senatori della 13ª Commissione - il Presidente, il relatore e tutti i commissari, della maggioranza e dell'opposizione - per aver avuto comprensione per questa situazione di difficoltà dalla quale partiva l'iniziativa del Governo e per aver prodotto il massimo sforzo possibile per un miglioramento del testo del decreto, senza fargli perdere quella efficacia operativa indispensabile che, se si perdesse, ne vanificherebbe totalmente la finalità. Credo che anche gli emendamenti apportati dalla Commissione più o meno concordemente (mi pare con una larga condivisione, almeno nella maggioranza dei casi) siano andati in questa direzione. Il dibattito in Aula ha altresì evidenziato dei punti di criticità anche di carattere generale, riferibili alla situazione dell'emergenza campana che, come è noto,

Io credo che, se il decreto può avere un merito, è proprio quello di fare una scelta coraggiosa, cioè quella di fissare un termine entro il quale il commissario delegato dovrà terminare le sue funzioni, e quella di prefigurare che cosa accadrà che sia finito il periodo dell'emergenza e, in qualche modo, ripristinato un contesto ordinario, anche di poteri e di responsabilità in capo alle istituzioni alle quali la legislazione ordinaria

la stessa norma finanziaria che è stata prevista, non quella che assiste gli interventi dell'emergenza, ma quella che deve sostenere la fase successiva dell'ordinarietà, cioè quella collegata al costo della tassa di smaltimento dei rifiuti regionale e che prefigura il rapporto tra

della Regione Campania; questo dopo averla nettamente distinta - com'è stato ricordato in un intervento molto lucido, al quale io rinvio, del senatore Morando, anche nella sua qualità

e che, evidentemente, se devono essere concluse entro il 31 dicembre 2007, non possono che essere coperte da risorse finanziarie già esistenti al 31 dicembre 2007 o comunque reperibili fino a tale data con il ricorso ai fondi disponibili della Protezione civile o degli interventi di emergenza. Se si tratta,

perché se non fosse quella la nostra interpretazione, dovremmo riconoscere che le misure contenute nel decreto-legge non sarebbero affrontabili con le risorse finanziarie

per esempio nel caso delle cave sottoposte a sequestro da parte della magistratura, dobbiamo riconoscere che la materia, ripresa, legittimamente, soprattutto nella pregiudiziale illustrata dal senatore D'Alì, ha trovato un esame ormai approfondito in tutte le varie sedi e istanze. L'Aula ha respinto la pregiudiziale di costituzionalità così motivata. Ma qui soprattutto mi piace richiamare l'intervento, molto preciso, del senatore Sinisi, che ha messo in evidenza la correlazione tra la utilizzabilità di beni sottoposti a sequestro e la ragione superiore che ispira questa utilizzazione, senza volere determinare alcuni elementi di conflitto con i poteri della magistratura o degli organi giurisdizionali, essendo più volte prevista nel nostro ordinamento la facoltà di utilizzare beni sequestrati, persino confiscati, anche senza un'ordinanza di requisizione. Qui

del commissario), non per capriccio ma per l'evidenziarsi di difficoltà impreviste lungo il cammino che si era proposto e che oggi lo costringono in qualche modo a navigare a vista, con un cronoprogramma di interventi

fino a pervenire allo smaltimento dei rifiuti che giacciono nelle strade o che non possono essere diversamente stoccati, e sino a quando non entreranno in funzione gli impianti, per così dire,

tra l'attività di smaltimento ordinario dei rifiuti e la loro destinazione finale), dico che lo sforzo che si sta tentando di fare con questo decreto-legge è proprio quello di tentare di ridurre questa contraddizione che è la causa non ultima - forse la principale - dell'aggravamento della situazione di emergenza in Campania. Qui non si tratta, allora, di compiere un atto di fede nei confronti del commissario; si tratta piuttosto una persona chiamata dallo Stato a svolgere una funzione delicata a realizzare tale funzione nell'interesse di tutti. Mi sarei immaginato e mi immagino che nel corso del nostro dibattito sugli emendamenti vengano indicazioni

siamo finiti. Consentirete dunque al rappresentante del Governo, che in questa sede ha la responsabilità di aver conferito una missione, una funzione tanto delicata al commissario,

si vuole assumere la responsabilità oggi di fare una ulteriore azione che non ci porti a conseguire quel risultato che tutti consideriamo indispensabile. Noi tutti non ne possiamo più della condizione di emergenza che c'è in Campania e tutti, se lo consentite, non ne possiamo più della necessità di affrontate questa situazione di emergenza con poteri straordinari, eccezionali, talvolta ai limiti della Costituzione, perché uno Stato non può sopportare a lungo che questo accada per una periodo che va al di là della ragionevole durata di una qualsiasi emergenza. Con questa motivazione, vi chiedo di aiutarci a convertire rapidamente e migliorare il decreto-legge, nell'auspicio che serva davvero a farci uscire da una condizione di gravissima difficoltà.

parere non ostativo presupposto che, come documentato dalla relazione tecnica, agli oneri aggiuntivi eventualmente sorti tra la data di entrata in vigore della norma relativa al differimento di un anno del periodo previsto per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 7, comma 1) ed il termine della dichiarazione dello stato di emergenza, si farà fronte con le risorse disponibili della gestione commissariale. Il parere è altresì reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 5 dell'articolo 1 vengano aggiunte infine le seguenti parole: "a valere sugli importi incassati con le tariffe di smaltimento"». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 9.0.1 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano in fine aggiunte le seguenti parole: "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per la partecipazione alle attività su indicate non vengono corrisposti compensi o emolumenti aggiuntivi.".

sui quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.50/2, 7.50/3, 7.50/4 e 2.32/1, mentre sull'emendamento 3.500 il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione delle parole: "Successivamente alla chiusura del sito saranno avviati gli interventi di bonifica". Esprime infine parere di nulla osta su tutte le restanti proposte emendative.»

vorrei ricordargli che sono otto mesi che il Commissario sta lavorando, secondo me senza alcun risultato, e noi, ad oggi, ci troviamo a convertire l'ennesimo decreto che estende poteri

possa non domandare se si fa il bene dei cittadini della Campania, quando si deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, pianificazione della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria. Se questo vuol dire andare incontro ai cittadini della Campania, sono molto preoccupato.

Presidente, ho ritenuto di non presentare un subemendamento, ma di

di polipropilene per non fargli prendere acqua, accumulati da qualche parte. Quando arriverà, se mai ci sarà, l'apertura del primo inceneritore o temovalorizzatore - chiamiamolo come vogliamo - difficilmente saranno utilizzabili così come sono (non CDR, ma spazzatura pressata) e

Ho molti amici che hanno fatto e stanno facendo i presidenti di Provincia, che sono consiglieri regionali e so che queste robe che avete descritto, e sulle quali sono perfettamente e personalmente d'accordo, sono di competenza del Comune, della Provincia e della Regione.

adottare un provvedimento centralista, secondo cui lo Stato obbliga una Regione a fare la raccolta differenziata in un certo modo perché la Regione, la Provincia e il Comune autonomamente non lo fanno? Spiegatemelo. Noi siamo padani e abbiamo subìto da decenni la colonizzazione culturale che non ha portato granché, se non una questione transitoria; però l'abbiamo avuta, per cui i nostri ragazzini magari hanno qualche deformazione mentale. Siccome da noi in casa il dialetto non lo parliamo più, ogni tanto viene qualcuno a parlare con l'accento siciliano o calabrese, visto il tentativo di deviazione culturale fin da bambini.

che, immagino, con questi padri fondatori a cosa darà origine? Perché non è qui a giustificarsi delle cose che ha fatto? Gli avete fatto fare anche il commissario straordinario per non so quanti anni. Avete speso in dieci anni 2 .000 miliardi di vecchie lire che anch'io e la mia famiglia abbiamo pagato, anche se a casa nostra facciamo il 60 per cento di raccolta differenziata. Avete assunto 2.000 spazzini in più, scortati dalle guardie del del Comune o dall'esercito, dalla Polizia o dai Carabinieri perché altrimenti gli sparano per strada, che si sono aggiunti ai 5.000-6.000 che esistevano già e che da quando sono arrivati questi non hanno fatto più la raccolta per le strade di Napoli e della Campania. Ma in che razza di paese siamo?

e poi in televisione sul satellitare vedono sedute come questa. Voi oggi nelle mie terre siete andati al 16 per cento, terzo partito, tutti insieme, rispetto ai partiti normali. Alla prossima tornata elettorale arriverete ad una certa cifra. Ma non fate poi il *tour* di Veltroni al Nord o la passeggiata in barcone sul Po. I rifiuti di Napoli da soli bastano a non farvi vincere in Settentrione e nella Padania per i prossimi cinquant'anni.

In tutta la provincia, con 850.000 abitanti che pagano le tasse, se facciamo in italiani equivalenti, di 3 milioni di italiani, abbiamo circa 800-850 persone addette alla sicurezza tra polizia e carabinieri,

la Patria italica ci ha regalato un bel pacco con dentro qualche migliaio di persone in soggiorno obbligato. Queste le fantasie

Fate gli studi di settore, ammazzate gli artigiani, ci mandate la Guardia di finanza in casa per controllare fino all'ultima vite che si dichiara nel bilancio come rimanenze finali e poi trovate i soldi per utilizzare mille persone per fare una cosa inutile!

se così non fosse, non saremo qua a discutere ed a parlare dell'emergenza rifiuti. Allora, se emergenza è, credo che l'emendamento 1.500/28, cari compagni, dovrebbe essere votato proprio per essere coerenti con quello che state dicendo. dicendo. Con questo emendamento diamo l'opportunità al commissario delegato di decidere caso per caso e in emergenza

Ecco perché sosteniamo che questi Comuni dovrebbero essere esclusi. Quindi, insistiamo sulla soppressione di tale individuazione delle discariche. Fermo rimane che è compito del commissario scegliere le discariche per affrontare l'emergenza

stimolare la riflessione dei colleghi. Ci si riempie tutti la bocca di parole come federalismo, enti locali, democrazia diretta, voce dei cittadini, eccetera. Non capisco allora perché siamo qui a decidere cosa devono fare nella Regione Campania, non solo dal punto vista dei soldi, di cui parleremo dopo e che comunque sono un aspetto importante, per ovvie ragioni, ma anche per situazioni così specificamente locali come l'individuazione dei siti. L'ho detto prima e lo ripeto: da tempo immemorabile queste terre sono governate della sinistra. Quindi, non sono perfettamente d'accordo sul fatto che i cittadini campani non abbiano nessuna responsabilità:

come si può pensare che possa essere il Senato della Repubblica a dire dove si può e dove non si può? Da decenni, lo ripeto ancora, la Campania in tutti i suoi territori è governata da amministratori locali di sinistra, quindi per definizione vicini al popolo; e all'interno di queste amministrazioni non mancano i Verdi, quindi persone in teoria particolarmente attente

Sulla questione della scelta: siete tutti comunisti, siete tutti compagni, governate da tanti anni quei territori e quindi non avete avuto problemi di Giunte uscenti di destra, di gente che vi ha fatto dispetti, che ha fatto piani regolatori. Vi siete gestiti tutto in famiglia; non so se a Napoli siete in famiglia come in altri territori, comunque il concetto è quello, vi siete gestiti tutto in famiglia. Ebbene, com'è possibile che oggi, dopo tanti anni, non sappiate neanche dove mettere quei

che poi da qualche parte devono essere messe. Quindi, esaurite le discariche e realizzati i termovalorizzatori, una discarica per gli inerti che arrivano dai termovalorizatori dovrete trovarla. Ebbene, tutte queste cose ovvie, che in tutte le altre regioni d'Italia si fanno, perché dove governate voi non ve le siete fatte?

Lira più, lira meno, negli ultimi dieci anni sono stati spesi 2.000 miliardi di vecchie lire (più di un miliardo di euro) in più rispetto a quella che era già la spesa normale degli enti locali e dei cittadini dello Stato, visto che la Campania riceve i fondi dallo Stato centrale per gestire in condizioni normali, routinarie, la spazzatura.

2.000 miliardi di vecchie lire tirati fuori dalle tasche di persone che magari prendono 450 euro al mese di pensione dopo 40 anni di attività lavorativa: glieli tirate fuori dalle tasche e li mettete in un bilancio dove (lo abbiamo visto l'anno scorso) ci sono 70.000 euro solo di telefonate su linee erotiche. Ma dov'è la magistratura? Arriva il Commissario straordinario e la prima cosa che fa è: segretaria, portaborse, auto blu, scorta. Ma dove siete? Dove siete?

della spazzatura e gli diamo l'ufficio, la segretaria, l'auto blu, l'autista e la guardia del corpo! Su queste cose nessuno ha niente da dire? Questo non è sperpero di denaro pubblico? Fate qualche riflessione.

in questi ultimi anni di legislatura... PRESIDENTE. No, è stata negata molte volte, presidente Schifani, lei lo sa perfettamente. SCHIFANI *(FI)*. La prego di farmi parlare; lei ha diritto di parola quando vuole presiedendo la seduta. La prego di essere un attimo più attento alle richieste dell'opposizione. Questa opposizione ha votato a favore di questo emendamento, ed essendovi degli scarti che ella conosce, la invito a fare a fare in modo che le votazioni elettroniche abbiano qualche secondo in più. In questo pomeriggio si sta infatti assistendo ad una compressione di qualche secondo sulla consuetudine del voto elettronico. Questo è un dato oggettivo

di attenersi, come ella è solito fare, al rispetto delle consuetudini del Senato, alle quali crediamo e delle quali lei è stato sempre rappresentante autorevole. Senatore Schifani, accolgo tutte le raccomandazioni, ma le posso assicurare che non sono il Vicepresidente più veloce del Senato; ce n'è uno che mi supera di gran lunga.

Dichiaro aperta la votazione.

voto favorevole in simpatia con il ministro Mastella, glielo dico francamente, perché, in casa del ministro Mastella si consumano, come in tutte le famiglie, dei drammi, qualche volta, e capita che le mogli abbiano pareri differenti rispetto ai mariti e che ci siano in qualche modo dei conflitti. Ebbene, voglio dare la mia testimonianza e la mia solidarietà al ministro Mastella perché mi sembra di ricordare che sulla medesima questione la sua gentile signora sia scesa in piazza contro la realizzazione del termovalorizzatore di Acerra

cercando di unire le due istanze, quelle governative e quelle dell'opposizione, perché molte volte questo Governo governa da una parte e poi fa opposizione:

Sì, signor Presidente. Non si capisce perché su competenze comunali debba intervenire addirittura il Ministero dell'ambiente: a competenze che abbiamo già assegnato dove è già presente il Governo per delega, perché c'è il commissario delegato. delegato. Qualcuno deve spiegarmi perché si deve ascoltare il Ministero dell'ambiente: forse per aumentare la confusione che c'è già e che state facendo, soprattutto per quel che riguarda la raccolta differenziata!

Forse qualcuno non se lo ricorda più che queste Province sono governante da quei rozzi leghisti? Non vorrete mica che i leghisti governino meglio di Bassolino! Non scherzeremo mica? C'è qualcosa che non va, sapete! *(Applausi dal Gruppo*

al Governo una pausa di riflessione, perché comprendo le motivazioni che portano alla riformulazione:

almeno nello spirito con cui abbiamo lavorato in Commissione, sia quella di rispettare l'area del Parco. Su questo punto chiederei se è possibile un accantonamento per fare una riflessione più compiuta e più serena e

Signor Presidente, ritengo personalmente che le modifiche apportate con approvazione di sub-emendamenti non possano più essere rimesse in discussione, e che quindi la riflessione che chiede il presidente Sodano può essere una riflessione d'approvazione o meno del testo di questo sub-emendamento, ma non può essere di ulteriore modifica; questo mi pare che sia chiaro. Non è che io sia contrario a questa riflessione, ma vorrei che il Governo ed il relatore si esprimessero sulla

all'Aula la differenza sostanziale che esiste tra queste due edizioni non guasterebbe, per l'intendimento di tutti), ma vorrei che si procedesse alla votazione, signor Presidente. Abbiamo già votato un subemendamento a questo emendamento, non credo si possa ulteriormente accantonare.

quindi della frazione cosiddetta organica. Questo emendamento, devo dire, veramente riassume tutta l'arroganza e la supponenza di quello che stiamo facendo. Nel mio Comune, tanto per avere un riferimento, che da quattro amministrazioni è governato da un sindaco leghista, e dove abbiamo superato il 60 per cento nella raccolta differenziata, facciamo ovviamente da anni anche la frazione organica; stiamo organizzando adesso la raccolta differenziata del vetro per colore, come fanno in Svizzera (probabilmente lo faremo fra qualche mese), prima, però, di arrivare a quella organica abbiamo percorso tutti gli scalini normali

che è la prima in assoluto, partita più di trenta anni fa, per un motivo molto semplice: che indipendentemente dalla volontà dei Comuni e delle amministrazioni, il vetro ha un contenuto energetico tale che la raccolta della bottiglia di vetro già fatto copre tutti i costi di raccolta, trasferimento

e quello quasi riesce a ripagarsi la raccolta differenziata. Anche in questo caso, non si guadagna tanto in peso, ma si guadagna moltissimo in volume e visto che la Campania non ha inceneritori, ma solo discariche, solo la raccolta delle bottiglie porterebbe via poco peso ma moltissimo volume e ovviamente le discariche sono dei buchi che si riempiono e si riempiono a volume e non a peso. Neanche questo viene fatto. Poi ci sono le raccolte che si fanno nei centri comunali: il legno, l'alluminio, il ferro, tutte cose che poi si aggiungono per strada. Per ultimo, quando veramente la sensibilità della cittadinanza è maturata negli anni, si fa anche la raccolta differenziata della frazione organica o umida, che effettivamente richiede una certa

per la raccolta differenziata della frazione organica da inertizzare per rimodellare la natura campana. Sono contento che ci sia questa previsione; sono anche d'accordo e personalmente la voterò, però sottolineiamo una volta di più veramente l'assurdità di un provvedimento che tralascia le cose importanti, non si interessa dei soldi, non si interessa degli sprechi, non si interessa delle responsabilità politiche, che sono enormi, e però ci dice come dobbiamo raccogliere quel 5‑6 per cento, se andrà bene, di frazione organica. Complimenti; siamo veramente alla fiera dell'inutile. Quello che serve non si fa da 30 anni, però ci preoccupiamo di raccogliere, forse tra 50, la frazione umida. Complimenti alla maggioranza e alla sua componente verde, soprattutto.

contrasta con un verbale firmato in prefettura da Bertolaso e anche con il buon lavoro della Commissione cui ha fatto riferimento il relatore.

Presidente, il Governo su questo punto si rimetterebbe all'Assemblea, nel senso che io non credo ci sia bisogno di un'ulteriore riflessione. Vorrei rassicurare il senatore Sodano corrisponde all'esigenza di pervenire gradualmente, come sarà indispensabile, alla utilizzazione della attuale materia trattata nei CDR in maniera tale che diventi diventi frazione organica stabilizzata. Ci sarà una fase iniziale nella quale questo avverrà gradualmente, brevissima, per la quale io non riterrei nemmeno di indicare un termine che potrebbe essere troppo lungo e che eventualmente sarà necessaria - non è nemmeno certo - per determinare invece la finalità che la Commissione indica come obiettivo di questa ulteriore destinazione del sito di Terzigno che è quella della esclusiva esclusiva ricomposizione morfologica del sito medesimo. Questo è l'obiettivo. Per renderlo possibile è necessario un momento di passaggio graduale dalla situazione esistente alla situazione diciamo a regime, che non è nemmeno a regime ma di immediata applicazione. Ecco la ragione per la quale non riterrei necessario questo approfondimento; così il Governo così il Governo interpreta l'emendamento che ha proposto. Se può bastare questo chiarimento, può far superare la richiesta di un accantonamento ai fini di una riflessione.

Siccome abbiamo scelto di non inserirla, perché era sbagliato tenere delle comunità in contrapposizione, potremmo mantenere i 60 giorni come limite massimo entro cui questa operazione, che veniva illustrata dal sottosegretario D'Andrea,

ancorché suscettibile di ulteriori interpretazioni, che in questa sede francamente non ci interessano da un punto di vista legislativo e normativo. Pertanto, sulla base delle dichiarazioni che sono state fatte, devo mettere ai voti l'emendamento della Commissione, integrato con la proposta

il motivo per cui la Commissione aveva utilizzato la dizione contenuta nell'emendamento 1.19, ossia rendere sostanzialmente inutilizzabile il sito di Terzigno, che si trova all'interno del Parco nazionale del Vesuvio. Le modifiche apportate, prima con l'approvazione del subemendamento, poi con la proposta del Governo, evidenziano la possibilità di un immediato uso. La parola "finale" introdotta dal Governo è chiaramente intesa nell'autorizzare nell'immediato un tipo di conferimento, mentre poi nella parte finale della sistemazione di quel

Va bene. Attiveremo i senatori segretari a fare in modo che ciascuno voti per sé, come sino a questo momento abbiamo fatto, senatore Boccia!

finestra"), riguardante l'Unità operativa complessa di ipertermia oncologica del Policlinico di Tor Vergata di Roma. Ho voluto sollecitare interrogazioni riguardanti gravi problemi sociali ed auspico che la Presidenza del Senato costringa davvero a rispondere un Governo che ritiene di non rispondere mai alle interrogazioni.

Grazie,